14.100 si prevede che nelle imprese confiscate o sequestrate l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice, assicuri la manutenzione ordinaria o straordinaria dei beni a lui affidati conferendo tali attività prioritariamente ad altre imprese confiscate. Ciò perché le imprese confiscate

ormai da due anni sono entrate in uso le nuove procedure per la risoluzione delle crisi bancarie, quindi sono stati introdotti meccanismi dai nomi ormai abbastanza tristemente noti come il *bail in*.

esse affrontano una situazione di crisi con una serie di specifiche, con una scaletta delle priorità e con alcune esclusioni. Da queste esclusioni ne mancano però alcune che sarebbero importanti: una - ad esempio - riguarda i conti che derivano da procedure fallimentari; un'altra esclusione importante è quella che proponiamo noi, e cioè escludere i conti dove affluiscono i beni sequestrati e confiscati. tratta chiaramente di una situazione limite che speriamo non si verifichi mai: nel momento in cui i beni confiscati affluiscono in un conto corrente (quindi il controvalore di questi beni), o conti o conti sequestrati affluiscono in un conto corrente di una banca che va incontro per qualche motivo a una procedura di risoluzione, quei conti sarebbero soggetti al *bail in*,

Mi permetto di suggerire, laddove non fosse possibile l'accoglimento come emendamento, che si valuti quanto meno da parte del Governo l'opportunità di

Signor Presidente, come ho già detto in discussione generale, ho ripresentato sotto forma di emendamento un disegno di legge depositato e fermo in Commissione affari costituzionali, in cui intervengo sulle misure di prevenzione personale,

di impedire ai sorvegliati speciali per mafia di fare campagna elettorale era limitato soltanto alla violazione della legge n. 212 del 1956, che riguarda l'affissione dei manifesti elettorali. Che io sappia, non ho mai visto in Calabria mafiosi attaccare Il tentativo che stiamo cercando di fare da quando è iniziata questa legislatura è riportare questo disegno di legge alla sua formulazione originaria, che prevedeva appunto una condotta specifica, dichiarando esattamente cos'è la campagna elettorale e impedendo ai sorvegliati speciali di fare campagna elettorale. In alcune zone della nostra Italia, soprattutto nel Sud, sappiamo perfettamente come si fa questo tipo di campagna elettorale. conosciamo le passeggiate che vengono fatte e i caffè che vengono offerti. Sono queste le manifestazioni attraverso cui la mafia mantiene per intero il suo predominio in alcune zone. Noi vogliamo che finalmente si impedisca

al Sottosegretario, anzi ai Sottosegretari, i Dioscuri, che ci stanno ascoltando, se è possibile almeno accettare la proposta nella forma attenuata di un ordine del giorno. Ricordo che nella storia degli atti parlamentari, quando fu approvata nel 2010 la formulazione dell'articolo 67, comma 7, fu approvato anche

Franco Roberti, che mi sembra di poter dire che viene ascoltato dalla maggioranza, in considerazione anche dell'emendamento approvato ieri. A dire la verità, Roberti dice anche altre cose,

richiamare le parole del procuratore Roberti per spiegare la *ratio* di questo emendamento: «Avevo «Avevo segnalato,» - sono parole di Roberti - «durante le numerose audizioni in Parlamento, una vera smagliatura nel sistema delle certificazioni antimafia. Parlo della norma in vigore nell'attuale codice che consente alle imprese mafiose di partecipare, dietro prestanome agli appalti pubblici come componenti dei consorzi stabili, eludendo la normativa e sfuggendo ai controlli con l'espediente di partecipare al consorzio in misura non superiore al 10 per cento». Ecco, questa è la smagliatura, ossia la possibilità di partecipare, per le società con interdittiva antimafia,

antimafia, in modo da bandire nella maniera più completa, totale e assoluta la possibilità, per le aziende che hanno un'interdittiva antimafia, di partecipare ai lavori pubblici sotto mentite spoglie, all'interno di un consorzio che vincesse una gara o un appalto pubblico.

È vero che dei passi in avanti sono stati fatti ed è stata svolta anche una discussione in Commissione rispetto al problema della conoscibilità e della conoscenza delle interdittive antimafia

la conoscibilità a livello nazionale della sussistenza dell'interdittiva, vanifichiamo qualsiasi sforzo che sosteniamo in questa direzione. Il mio appello è rivolto al Governo, visto che è in

le lacune presenti oggi sul territorio nazionale e che comportano i ritardi nella conoscibilità e nella conoscenza della sussistenza delle interdittive antimafia sul territorio nazionale.

Quali sono le motivazioni? Secondo me dovrebbe essere il contrario: più presidi istituzionali sono presenti in certe città, più si accresce la fiducia della gente nello Stato e in quanto esso rappresenta.

molto più rispondente alle finalità della legge istitutiva. Tuttavia, l'idea originaria era sostenuta dalla consapevolezza che occorreva avere avere persone con professionalità - già possedute o da acquisire - tali da poter essere garantite attraverso qualità personali degli operatori all'interno dell'Agenzia. Per tale ragione, la quantità delle sedi aveva portato a individuare un numero di 200 dipendenti

e l'altra metà ricorrendo alla mobilità. Cos'è avvenuto? La Commissione bilancio, correttamente, ha posto in evidenza che quel sistema non era tale da poter essere garantito con la copertura già prevista. E, quindi, si è pensato di prendere tutte le 200 unità con la mobilità. ha esperienza come me della mobilità che è stata attuata in alcuni uffici giudiziari e qual è stato il risultato. Mi sono chiesto, quindi: è proprio necessario? Siccome l'utilizzazione di più sedi non è funzionale ai compiti dell'Agenzia, rendiamo l'Agenzia effettivamente funzionale lasciando due sedi,

il numero delle sedi deve necessariamente essere ridotto, perché la frammentazione dei comportamenti degli appartenenti all'Agenzia a seconda delle sedi non è tale

sono illustrate e specificate con l'emendamento 27.108, che tutti voi potete valutare e apprezzare. Si tratta di valorizzare. Non parlate di professionalità e di merito quando poi fate delle scelte basate sulla mobilità.

Signor Presidente, la leggerezza con cui si affronta questo voto mi lascia assolutamente perplesso. La conferma in Aula del presidente Tonini del

inoltre non hanno neppure gli stessi criteri di indipendenza e autonomia di professionisti che possono essere selezionati esattamente per queste funzioni in ragione della loro esperienza e delle loro competenze tecniche. Il timore del Movimento 5 Stelle è che si vada a concedere ad un vero e proprio carrozzone pubblico, che si è anche caratterizzato per fatti molto gravi negli ultimi anni, una responsabilità veramente rilevante come quella della futura gestione delle società più importanti che vengono confiscate alla malavita organizzata. qualche risultato, perché si è affiancata alla possibilità di nominare un amministratore giudiziario dipendente di Invitalia anche la possibilità di nomina di dipendenti dell'Agenzia per la confisca. Questo, a nostro parere, è un passo in avanti

era solo un mio possibile convincimento, non una certezza e non essendo una certezza non era giustificato il modo in cui sono intervenuto. Il mio è un atteggiamento garantista,

dottrina ampiamente dibattuta anche a livello europeo (ci sono stati diversi ricorsi e sentenze successive da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo), in ultimo rinnovata anche per la legge sui *foreign fighter.* Sappiamo

quanto riguarda la proporzionalità, in questo caso il punto centrale di tutta la dottrina è se la compressione del diritto soggettivo può essere bilanciata dall'interesse collettivo.

tutto perché stiamo introducendo la possibilità del sequestro nel caso in cui si parli di associazione a delinquere. Ma io, nella mia breve esperienza di paragiudice della Giunta per le autorizzazioni a procedere, non ho mai visto casi di corruzione che non siano in forma associativa.

Ecco il perché della mia animosità di ieri, perché quello che sta succedendo mi sembra un appesantimento del diritto penale in Italia se prima abbiamo parlato, nei casi di terrorismo o di associazioni criminali, di necessità e proporzionalità esistenti, adesso che stiamo parlando di corruzione, chi potrebbe impedire che un giorno, sulla base di questo precedente, non si parli di necessità anche per la tutela ambientale per i reati sui minori? Capite bene che dall'eccezionalità passeremmo alla normalità e normalità, in questo caso, significherebbe uno Stato in cui la possibilità requirente diventa così potente il passo verso uno Stato di polizia - non gridate allo scandalo, è chiaro che io esalto ed esaspero il dibattito per far capire quale decisione stiamo prendendo - sarebbe Non possiamo poi ridurci ad auspicare un intervento della Corte costituzionale, del Capo dello Stato o della Corte dei diritti dell'uomo. La prima responsabilità è nostra, è cercare di capire quello che stiamo facendo e se davvero la necessità e la proporzionalità sono tali da poter assumere decisioni così gravi. Ecco il motivo, Presidente - e continuo a chiedere scusa dei miei eccessi di ieri - per cui continuerò a votare contro

di particolare interesse, anche sotto il profilo del numero dei dipendenti, cioè quelle aziende per le quali è ammessa la procedura straordinaria ex legge Prodi

delle spese dello Stato perché, chiaramente, i compensi degli amministratori giudiziari per le grandi aziende sono notevoli e in questo caso è previsto che l'amministratore giudiziario indicato da Invitalia continui a percepire gli emolumenti che gli vengono dalla sua posizione di dipendente di Invitalia e non per le attività di amministratore giudiziario, salvo ovviamente il recupero delle spese per le attività di amministrazione.

tutto questo corretto, anche se è distonico rispetto alla previsione dell'amministratore giudiziario nominato nell'ambito di una procedura di interdittiva

perché in odore di mafia non può svolgere alcuna attività di straordinaria amministrazione quale, per esempio, quella di dare continuità all'azienda attraverso la partecipazione a gare pubbliche. Quando invece invece il sequestro avviene nell'ambito della procedura per le misure di prevenzione, tutto questo può essere fatto dall'amministratore. Notate la distonia? Vi rendete conto che, a questo punto, è preferibile per l'imprenditore subire un sequestro nell'ambito delle misure di prevenzione piuttosto che subire un'interdittiva antimafia?

Quando mi sono reso conto che il testo base non prevedeva l'inclusione di quelle regole che avevo immaginato nell'ambito delle interdittive antimafia, ho presentato degli emendamenti

di questa parte del codice antimafia che lascia fuori dalla porta una materia che ha fatto molto rumore, inducendo anche qualche magistrato ad iscrivere nel registro degli indagati un nostro collega,

Credo di averla sistemata bene, però non mi sono mai state dette da alcuno le ragioni per cui questa materia è rimasta fuori dalla porta e non si è data la possibilità di includerla nel codice antimafia, cosa a mio avviso

che attengono anche alla possibilità di un aumento delle aziende e imprese che rientrano nella *white* *list*,

di parole che servono a declamare una volontà di legalità e un modo di essere della nostra azione contro la corruzione quando cui si tratta di intervenire con strumenti chiari e precisi per allargare il tasso di legalità si vota contro. Queste sono le cose più assurde.

non l'avevo pensato, lo riconosco, ma lei sa meglio di me che quando lavorammo al codice antimafia la questione fu dibattuta a lungo. c'erano problemi di struttura delle prime azioni di *rating*. Mi domando, pertanto, perché oggi non possiamo ampliare quest'ambito. Ero convinto che avremmo trovato la soluzione. Certo, non facendo parte della maggioranza già è tanto se molte volte sono riuscito a dare un contributo a migliorare il testo,

non prevedeva questo obbligo, ma, nell'ambito delle attività di manutenzione, introduceva e introduce la priorità per le imprese fornitrici.

si preferiscono le imprese fornitrici di lavoro già sequestrate ovvero confiscate. Siccome qui ci stiamo occupando di queste aziende, sembra una bella cosa perché diamo una mano ad aziende che, come è stato detto, sono spesso in difficoltà.

una è stata oggetto di sequestro e l'altra no. Chi scegliamo per fare la manutenzione? L'azienda che è stata già sequestrata o confiscata.

i servizi di quell'azienda, l'azienda che sceglie questi servizi intanto è meno competitiva, avrà introiti inferiori, spese superiori, senza contare che esistono anche - grazie al cielo - le aziende che non sono sequestrate o confiscate, che si sentono dire che la loro offerta era la migliore,

si limitano a guardare il problema, dimenticando che esiste anche un altro mondo, il mondo delle aziende non sequestrate, il mondo reale dove l'economia deve tenere altrimenti

rilevando che nella generalità dei casi le aziende a conduzione mafiosa hanno anche un tessuto interno di quella derivazione.

l'amministratore preferisca utilizzare quel servizio ed affidare quelle attività ad altra impresa confiscata.

per l'azienda che la richiede. Io ho delle perplessità, a meno che questa non sia una prova tecnica di laboratorio di nuove maggioranze politiche; ma su questi argomenti io credo che la politica - così come stiamo dimostrando io e i miei amici di Gruppo - deve rimanere fuori dalla porta. Sono materie delicate che vanno trattate

il giudice delegato e l'amministratore giudiziario hanno tutta la discrezionalità per decidere se affidare il lavoro di manutenzione a un'impresa di mercato o a un'impresa sequestrata o confiscata.

(istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate). Sempre con il nobile e condivisibile fine di

Questo tavolo cosa fa? Favorisce la continuazione dell'attività produttiva; dà ausilio all'amministratore con dei buoni consigli, a quanto pare. Favorisce la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate Favorisce la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate nel percorso di emersione alla legalità (questo è mica male, ci mancherebbe che non dovessero emergere alla legalità); Il tavolo provinciale è composto dal meglio che abbiamo: un rappresentante dell'Agenzia, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un

istituiti quando è troppo tardi e, ahimè, possono tutt'al più favorire l'intervento degli ammortizzatori sociali per i lavoratori che si trovano senza più il datore di lavoro, ma non molto oltre questo. mi chiedo se non avete mai sentito parlare di aziende che si trovano in difficoltà per motivi diversi dal fatto di essere state sequestrate per mafia. E allora perché a queste che sono state sequestrate per mafia diamo l'ausilio di tutte queste fulgide menti, sicuramente nominate in questi tavoli a costo zero, senza il rimborso di un centesimo? Ciò peraltro vuol dire che, anziché fare altre cose (perché si suppone che il loro lavoro sia anche utile), devono fare questo. Quando si dice senza ulteriori oneri vuol dire che, con i mezzi che ci sono oggi per fare altro, gli facciamo fare queste cose. Ne consegue che le aziende che sono in difficoltà perché sotto sequestro per questioni di mafia hanno il supporto di tutti questi signori;

per fare in modo che persone responsabili ed esperte, quali si suppone siano tutti i componenti del tavolo, si trovino e diano una mano o un consiglio, a maggior ragione per emergere alla legalità. Se è solo per riempire con un ulteriore articolo una legge, forse una legge è più efficace, è più leggibile e produce migliori effetti se è composta solo dalle parti utili, non con un tavolo a costo e a effetto zero, che, se funziona, crea una situazione di favore ad alcune aziende rispetto ad altre, i cui dipendenti non hanno nulla di meno rispetto ai dipendenti di un'azienda confiscata per mafia.

forse anche i suoi dipendenti potrebbero avere qualche collegamento, a meno che io apprenda ora che le aziende mafiose effettuano le loro assunzioni attraverso rigorosi concorsi.

«Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, sentito il competente tavolo provinciale permanente di cui all'articolo 41-*ter*, previa autorizzazione del giudice delegato, e l'Agenzia possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini a quelli in cui opera l'azienda sequestrata o non definitivamente confiscata». Questa differenza non la comprendo; non capisco l'ausilio che può dare un'azienda concorrente sul territorio per la crescita dell'azienda confiscata, ma qui stiamo Continuo la lettura: 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prescindendo dai limiti di fatturato, individuati nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, attraverso procedura ad evidenza pubblica - quali sarebbero? Non indette dall'amministratore giudiziario, tenendo conto dei progetti di affiancamento dagli stessi presentati e dell'idoneità a fornire il necessario sostegno all'azienda». Se qualcuno in questa Assemblea mi dice di aver compreso ciò che ho letto, io mi confronto nel merito. Poiché però credo che, non avendo capito io che non sono tra i più stupidi di questo Senato

così come rimarrà, perché voi siete sordi ai suggerimenti tecnici, ma anche letterali - se mi consentite - noi non lo votiamo.

Costituzione, lo ritiriamo con molto rammarico, perché trattava della concessione degli immobili al personale delle forze di polizia, delle Forze armate

Signor Presidente, senza alcuna vena polemica, probabilmente il dispositivo, in maniera casuale, a volte lascia un frangente di tempo in più. Le assicuro che questa volta la verifica si è chiusa subito; probabilmente c'è stato un malfunzionamento. Non so. «L'operazione di registrazione dei richiedenti viene attivata dal pannello di comando del Presidente e deve essere effettuata dai senatori entro il termine di cinque secondi. Coloro che intendono Coloro che intendono appoggiare la richiesta di verifica del numero legale o di votazione qualificata devono introdurre…» e segue per queste operazioni c'è un termine, da Regolamento, di cinque secondi, scattato il quale l'apparato blocca le votazioni.

di come noi, a parole, diciamo di voler dare testimonianza dell'attenzione che portiamo al lavoro e al sacrificio Io ho presentato l'emendamento 18.0.100,

«dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Avendo ricevuto parere contrario dal bilancio, i relatori, probabilmente distratti,

il povero cristo poliziotto che va in un'altra città, lontano dalla sua casa e dalla sua famiglia, deve pagare l'affitto - questo c'è scritto -

quindi non potete continuare con questo giochino di affermazioni verbali non seguite da comportamenti conseguenti. Leggetelo, vi prego: non c'è una spesa!

Presidente, con l'emendamento 18.0.102 avevamo inteso riproporre un *modus operandi* che era stato riconosciuto efficace e molto importante nel contrasto alle agromafie. Abbiamo ripreso il protocollo di legalità

dopo l'incontro in Commissione antimafia eravamo tutti d'accordo che quella misura dovesse diventare addirittura un atto avente forza di legge, in modo tale da farlo diventare un *modus operandi* di tutte le amministrazioni che gestiscono questa tipologia di beni.

adesso c'è un parere negativo. Vorremmo capire per quale motivo non va più bene questo *modus operandi*.

Voglio tranquillizzare l'Assemblea rispetto al fatto che su questo emendamento, oltre al limite strutturale che ci viene consegnato dalla Commissione bilancio, ai contenuti. Il protocollo, che - come sapete - è un meccanismo normativo secondario che serve a sperimentare strade nuove ad aprire nuovi percorsi e che ha un carattere pattizio tra enti viene di fatto disciplinato in una serie di norme già contenute all'interno del Testo unico antimafia. infatti, inserito il reato di truffa aggravata all'interno del novero dei reati su cui si può esercitare la misura di prevenzione patrimoniale

visto che nel dispositivo di tale ordine del giorno si chiede proprio l'attuazione delle legge Lazzati, cosa che condividiamo pienamente.

22.0.100 è stato ritirato.

mi domando se chi ha redatto il testo di questo articolo abbia mai avuto un minimo di esperienza nei tribunali di procedure fallimentari. di prevedere che il bene sottoposto a misura di prevenzione - e quindi a sequestro o confisca - non possa essere inserito nella massa

il bene sottoposto a sequestro praticamente non può essere aggredito. La confusione sorge però, in maniera ancora più palese, sotto il profilo procedurale:

per una ragione qualsiasi, la confisca o il sequestro debbano essere revocati e l'imprenditore ritorni nel possesso del bene sequestrato o confiscato, si riapre la procedura fallimentare. voi aprite e chiudete le procedure fallimentari e i procedimenti giudiziari con una certa facilità. Probabilmente scriverlo è facile, ma viverlo nei tribunali

che possono far capire se un creditore è una persona perbene, che ha impegnato i propri capitali in credito, fornendo servizi o beni strumentali.

perché credo che la coerenza vada sempre mantenuta, indipendentemente dalla politica. Io voterò a favore per tutto quello che ho detto nei giorni

Quale coerenza c'è da parte di chi, solo per disciplina di partito o di Gruppo, vota norme contrarie alla propria coscienza?

riprende interamente il contenuto dell'emendamento 24.0.100,

vuole procedere non soltanto senza coinvolgere il Parlamento, ma addirittura apertamente contro l'articolo 178

pignoli, gli zelanti, sui 50.000 euro o sui 150.000 euro, ma quando si tratta di un'opera che dichiaratamente costa 4 miliardi e che verrebbe compensata con 24 miliardi (mi riferisco alla Gronda di Ponente a Genova) va tutto bene. C'è una legge che dice che non si può fare e che non si possono fare proroghe, invece viene fatta una proroga che rende circa 10 miliardi di euro, in cambio di un'opera di 4 miliardi di euro. A questo si aggiunge un aumento dei pedaggi di altri 14 miliardi di euro e si arriva a 24 miliardi per un'opera da 4 miliardi; il tutto fatto alla luce del sole. Ma su questo, silenzio assoluto. Anzi, leggiamo sui suddetti giornali che il Governo manda i suoi collaboratori a Bruxelles per perorare la causa, per andare contro una legge

Ci occupiamo, quindi, dei 50.000 euro con grande rigore e poi, quando si parla di 20 miliardi regalati a una società privata che già ha degli utili spaventosi, credo pari solo alle

per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, per le società cooperative,

26.0.301 i relatori vanno ad ampliare l'ambito di applicazione della norma che prevede l'informativa antimafia da parte di determinati soggetti. che anche gli imprenditori agricoli che occupano un certo numero di dipendenti debbano munirsi, in caso di richiesta di fondi europei, dell'informativa antimafia. Quindi si interviene in materia di informativa antimafia, quella stessa materia che il Presidente della Commissione giustizia ha deciso di non voler trattare in questo provvedimento, dichiarando i relativi emendamenti inammissibili. diversità di opinione rispetto alla materia non la comprendo. Ma, in ogni caso, l'esperienza ci insegna che per alcune imprese basta avere due dipendenti che hanno rapporti con la criminalità organizzata per avere l'interdittiva antimafia. Immaginiamo il caso di un imprenditore agricolo che assume stagionalmente dei dipendenti che lavorano nel fondo e che per caso si trova ad avere, tra questi lavoratori stagionali,

non ha la liberatoria antimafia. Ma non era il caso, presidente D'Ascola, Governo, relatori, di trattare la materia e di inserirla in maniera organica in questo codice antimafia? Io non comprendo perché: perché: c'era fretta? Vi ricordo che la fretta non è mai foriera di provvedimenti giusti, nell'interesse del Paese e degli italiani. sulla base delle mie personali convinzioni in tema di interdittiva antimafia, io non lo posso votare. Trovo giusto che si faccia la lotta alla criminalità, ma - come diceva ieri anche

accelerare l'approvazione di questo testo, non curandovi degli enormi errori che sono stati commessi sia sotto il profilo sostanziale, che sotto il profilo sistematico delle norme del nostro ordinamento.

come gli altri che ho svolto in Commissione antimafia, in Aula e in Commissione giustizia, sarà attenzionato in informative di Polizia, fornito a pubblici ministeri e anche utilizzato per dimostrare che chi ha idee diverse da quelle di alcune procure di per se stesso è un "erosore" di legalità o, peggio, uno che vuole favorire la criminalità. Noi ci siamo posti invece, con il senatore Falanga, un problema gigantesco, che continuo a riproporre

salvo poi scoprire che tutto è costruito su informative di Polizia, senza alcuna verifica seria e secondo le politiche delle prefetture, ognuna delle quali va per conto suo. Quindi, pur sapendo che la materia è delicata, ho chiesto con forza in Commissione che questo nodo venisse sciolto in Parlamento, cioè che si approfittasse

Ricordo ancora una volta che le interdittive antimafia - lo dico al Parlamento, ma lo ripeterò nelle dichiarazioni di voto finale su questo provvedimento e sui provvedimenti cautelari - sono basate sul «non si può escludere». La sostanza è che vengono date le interdittive e viene preclusa l'iscrizione alla *white list* delle aziende sulla base di presunzioni sintomatiche, che prescindono da qualsiasi reato o atteggiamento penalmente perseguibile e che attengono, non si può escludere che le parentele, le frequentazioni e i verbali che vengono prospettati indichino un pericolo futuro ed eventuale di infiltrazione. Siamo arrivati ad autorizzare

quando vivo situazioni di questo genere. Poteva essere l'occasione per parlarne, ma c'è stato detto di no e che non era il contesto; adesso però ritrovo emendamenti che trattano il tema dell'interdittiva. Spero che in questa legislatura, seguendo anche alcuni autorevoli suggerimenti del dottor Gratteri e del dottor Cantone, si possa arrivare a determinare una qualche garanzia giurisdizionale oppure si possa arrivare a tre prefetti anziani anziani esperti nella materia che possono coordinare le prefetture per evitare che il prefetto di una città faccia esattamente il contrario di quello di un'altra e che si resti in mano all'arbitrio assoluto in tematiche che costano il posto di lavoro a centinaia o migliaia di persone (salvo poi accorgersi che l'interdittiva era sbagliata). Mi associo al collega Falanga in questo rammarico. Magari manderò io direttamente alla procura quanto ho detto senza fargli fare la fatica di raccogliere quanto detto facendo il mio dovere di parlamentare, ovvero esprimendo le mie opinioni e dando i voti che ritengo più opportuni nell'interesse del Paese, con il rammarico che, per questa materia, non si sia approfittato di questo meccanismo per portarla almeno a essere conforme ai princìpi della nostra Costituzione.

all'Agenzia determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia medesima».

L'Agenzia attualmente ha 30 dipendenti, che hanno una certa professionalità ormai. Dico ai relatori: non dite che

Presidente Tonini,

voi la responsabilità, se fate fallire l'istituzione di una professionalità forte nell'Agenzia. Questo è l'ultimo passaggio. È evidente,

Nel 2011 io fui costretto, nella sede del Ministero dell'interno, ad accettare di mettere la sede principale a Reggio Calabria perché in quel momento bisognava inviare un segnale d'immagine.

Questa è la logica. È necessario un minimo di responsabilità e di volontà del Governo. Trovare la copertura per venti posti da mettere a concorso è veramente un'inezia, sottosegretario Migliore. Signor ministro Orlando, mi affido a lei. Si tratta di trovare soldi per coprire venti posti da mettere a concorso per l'Agenzia. Se vogliamo avere del personale qualificato, trenta unità ci sono già e, quindi, con una piccola riformulazione da parte dei relatori, possiamo arrivare ad avere un sistema coerente con le finalità che ci poniamo. a sostegno della richiesta del senatore Caliendo di accantonare l'emendamento per consentire una ulteriore riflessione ai relatori e al Governo, io segnalo una distonia nell'ambito dell'articolo 27. 27. Con l'articolo 27, infatti, viene affermata la personalità giuridica di diritto pubblico dell'Agenzia. Viene detto espressamente che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e personalità giuridica di diritto pubblico. Poi, però, i relatori prevedono con l'emendamento 27.301 il potere, attribuito al direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1, di stipulare contratti a tempo determinato al fine di assicurare

perché, tra le vittime vere della mafia e di tutto ciò che gravita intorno, ci sono i testimoni di giustizia che spesso affrontano disagi gravissimi - il che a volte è un eufemismo, perché alcuni di essi sono stati anche ammazzati

l'impegno che finirà come gli altri - si chiede di estendere queste misure anche alle persone sottoposte a speciale programma di protezione che intendano mantenere la propria residenza o domicilio. Anche queste persone hanno bisogno di sostegno; anzi, a volte ne hanno bisogno più delle altre. Costoro non affrontano il grave disagio di spostarsi in luoghi molto diversi da quelli in cui hanno sempre risieduto,

ma in un provvedimento che è all'esame da più di un anno e mezzo non si è trovato il modo di reperire 10 milioni, quando per molte altre cose le risorse si trovano eccome, tra l'altro rapidamente e senza problemi,

anche che non si possa fare. «Pazienza, andiamo avanti. L'importante è andare avanti e dare il segnale al Paese»: dare il segnale al Paese che sarebbe giusto aiutare chi lotta contro la mafia in prima persona, esponendosi e rischiando la propria pelle e quella dei propri familiari, il proprio patrimonio e la propria attività,

che in Commissione giustizia del Senato si sta esaminando un disegno di legge per una riforma organica sui testimoni di giustizia,

presenti tutti i contenuti degli emendamenti in esame, che vanno a migliorare la condizione dei testimoni di giustizia secondo le indicazioni della Commissione antimafia, che ha compiuto un lavoro specifico su questo importante problema.

Insomma, siamo di fronte a un articolo ingarbugliato e vago e ripeto che le esperienze di applicazione delle deleghe sono state numerose e molto spesso del tutto negative: nella delega si dice una cosa e altra cosa fa il Governo. E, nell'ambito della giustizia, potrei ricordare la riforma della geografia giudiziaria, cui sia era dato mandato al Governo di fare una scelta di sedi giudiziarie e il Governo ha fatto uno sterminio. un partito, il partito maggioritario in quest'Aula e nel Parlamento in generale, si è presentato alle elezioni includendo nel proprio programma nazionale il ripristino di sei tribunali che erano stati cancellati:

è titolare del Ministero della giustizia, a emendamenti che rientravano nel suo programma elettorale nazionale ha votato contro. il Governo prima ha respinto i pareri dati quasi all'unanimità sia dalla Camera, sia dal Senato e, dopo aver detto ad essi di no, li ha messi nel proprio programma elettorale e di nuovo ha detto di no quando ha avuto direttamente in mano

imprenditori che prestano il loro servizio gratuito a favore delle aziende sequestrate o confiscate. Si sta veramente facendo un pasticcio. Questo articolo è forse un pasticcio peggiore degli altri, meritevole dunque di uno dei nostri pochissimi emendamenti. Se avessimo voluto fare un'azione per allungare i tempi, avremmo ben potuto presentare, senza difficoltà, moltissimi emendamenti. Ci si è contenuti al massimo, ma a quei pochi emendamenti viene detto di no,

spiegare il perché. L'unico perché è che vi ordinano di votare in un certo modo: direi che è davvero un perché molto piccolo di fronte a questioni serie come quelle che stiamo affrontando.

con la delega al Governo ad intervenire (peraltro entro quattro mesi) - sono qui presenti il ministro Orlando e il Sottosegretario: non so se hanno compreso che il tempo loro assegnato è di solo quattro mesi per emanare provvedimenti che regolamentino una miriade di materie che, peraltro, nella delega non vengono neanche puntualmente precisate.

tra quattro mesi, quando sarà eventualmente chiesta una proroga, perché i tempi tecnici e materiali per intervenire in una materia così ampia non ci sono.

Presidente, pur condividendo le motivazioni per le quali si voleva sopprimere l'articolo 32, e non essendo stato possibile proseguire su questa strada, credo che migliorare l'articolo stesso sia assolutamente un dovere. Troppo spesso le imprese che vengono sequestrate

i fornitori, lasciandole di fatto come delle scatole vuote. Peraltro, agli imprenditori che viene chiesto un tutoraggio gratuito, a volte viene creato un vuoto circostante mettendo addirittura in seria difficoltà le loro imprese. occorra sostenere questa attività gratuita, che è fatta non solo ed esclusivamente da tecnicismi, ma anche dalla passione e dalle competenze delle persone, prevedendo anche per le aziende degli imprenditori che prestano la loro attività in maniera gratuita delle forme di premialità fiscale e contributiva.

celare la realtà oggi consolidata che il sequestro di un'impresa faccia nient'altro che poi

produttività degli imprenditori e, di conseguenza, del Paese, un supporto tecnico sia dovuto e molto utile.

per di più, verosimilmente in un periodo di transizione tra una legislatura e l'altra. Non riteniamo pertanto prudente, in questo momento, dare una delega al Governo su materie di questo genere, con un con un ampio criterio di discrezionalità nell'eseguirla. Come ho già detto, sono numerosi gli esempi grazie.

Quando si dice che si deve fare una selezione delle sedi giudiziarie e poi si aboliscono tutte, tranne quelle espressamente previste da conservare nella delega, è evidente che il Governo non ha fatto alcuna selezione, per cui è già andato contro la delega.

tribunali, nel proprio programma di Governo. Ma tutte le volte che sono stati da me presentati degli emendamenti per ripristinare quei tribunali, copiando le parole del programma del Partito Democratico, il Governo ha detto di no, ivi incluso da quando è guidato dal ministro Orlando, esponente del Partito Democratico. Questa è una coerenza che ritengo lodevole e di cui gli elettori si ricorderanno: gli elettori che hanno votato anche perché nel programma era previsto quel punto, di fronte alla ripetuta bocciatura se ne ricorderanno. E ce ne ricordiamo anche noi e, quindi, prima di dare una delega ci andiamo piano. Ricordo una delega della fine della scorsa legislatura, sempre in ambito di giustizia, che prevedeva una riforma sulla questione della filiazione. votata dal Parlamento si chiedeva al Governo di formare il concetto di responsabilità genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potestà genitoriale.

È questo un modo onesto di esercitare una delega? No davvero. Il risultato è che con quel provvedimento lo Stato ha detto il potere è suo su tutti i bambini di questo Paese, e non dei genitori. La parola «potestà», che mai il Governo ha chiesto di abrogare, viene abrogata per decisione del Governo stesso, con un decreto legislativo che viola la delega. Vogliamo dare allora altre deleghe al Governo perché ne faccia lo stesso uso? No, grazie. Ci hanno già rubato i tribunali. hanno già rubato i tribunali. Non esiste più la potestà genitoriale, ma esiste la responsabilità: è come dire che il proprietario dei bambini, il padrone dei bambini è lo Stato. I genitori sono responsabili,

in un periodo in cui proprio questo Governo le ha violate in modo così spudorato, continuativo e determinato. Ora basta. Per cui "no" a questa delega. Ricordo inoltre che la delega non viene dall'opposizione, ma dalla maggioranza, che poi si trova nella condizione di non poter influire. Quei provvedimenti sui tribunali a cui ho fatto riferimento venivano contrastati anche dalla maggioranza, altrimenti non si sarebbe ottenuta la grande maggioranza parlamentare in alcuni casi l'unanimità, in Commissione giustizia sia alla Camera che al Senato. Eppure, è la maggioranza che si priva della possibilità di decidere. Voi della maggioranza potreste influire, ma rinunciate a influire, ben sapendo e avendo chiara l'esperienza

Auguri. Però anche gli elettori si ricorderanno di questi atteggiamenti.

le chiederei, prima di arrivare alla fine, di sospendere la seduta per dieci minuti, affinché i relatori possano determinare una correzione,

che un'indicazione di voto data dai relatori su un emendamento importante, su cui questa Assemblea si è già espressa, sia stata errata. Quindi ci potrebbe essere stato un errore materiale da parte della maggioranza, del Governo e dei relatori rispetto a un voto su un argomento che invece è assolutamente importante e prioritario.

e, rivolgendosi alla Presidenza, chiedesse l'annullamento e la ripetizione del voto di un emendamento. Signor Presidente, credo che il riferimento sia a un emendamento aggiuntivo all'articolo 30. Ieri avevo sollecitato un rinvio ad oggi della discussione, proprio perché vi fosse la certezza e la precisione degli emendamenti e dei pareri sugli stessi. Si è voluto proseguire non è stato ascoltato il mio consiglio. Credo di poter confermare quello che ha detto il senatore Cappelletti, che però si scontra completamente con quello che prevede il nostro Regolamento. In caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare e dispone l'immediata rinnovazione, con o senza procedimento elettronico. Noi abbiamo votato l'articolo 30 e - a memoria - il successivo articolo 32. In questo caso non c'è stata un'irregolarità di votazione; il relatore può essersi sbagliato su questo emendamento come su altri 80. Non lo so, però il parere era stato espresso, il Senato ha votato e non può tornare a votare nuovamente una cosa su cui si è già espresso.

Presidente, pensiamo di chiedere una sospensione e il rinvio della votazione degli ultimi articoli a martedì.

Presidente, facendo seguito a una richiesta già espressa precedentemente dal relatore chiedo che la fase della votazione degli emendamenti, che è pressoché conclusa, si interrompa in questo momento.

ne ricordo i nomi - Adele Puglisi, Claudia Maria D'Antona, Claudio Cappelli, Cristian Rossi, Marco Tondat, Maria Rivoli, Nadia Benedetti, Simona Monti e Vincenzo D'Allestro,

altro che non essere stati in grado di recitare versetti del Corano, e quindi di essere riconosciuti come estranei a quella religione. Lo voglio ricordare perché su quel terribile episodio è calata una cortina di silenzio

Devo sottolineare qui in Senato che, mentre, giustamente, l'Italia si è mobilitata, in tutti i municipi e nelle università, perché venga fatta piena luce sulla morte di Giulio Regeni, stranamente sulla morte di questi nostri nove connazionali è scesa una cortina di silenzio. Ebbene, credo non sia giusto. Credo sia giusto raccogliere il grido di protesta e di dolore dei loro familiari perché quello che l'Italia fa per altre persone, che sono state vittime di altrettanti gesti di violenza, possa avvenire anche per ricordare queste nove vittime del lavoro: erano italiani che lavoravano all'estero, vittime di una barbarie terroristica senza alcuna giustificazione. la ricerca della verità dei parenti di queste vittime che chiedono un minimo di appoggio del Governo italiano e del Ministero degli affari esteri, perché perlomeno vengano restituiti

perché questo avvenimento così tragico non passi sotto silenzio e venga fatta piena luce sull'accaduto. Mi sembrava importante, alla vigilia di questo accadimento, ricordarlo qui in Senato e ricordare i sacrifici di questi nostri lavoratori.

Signora Presidente, da mesi al Senato ricordiamo con interventi di fine seduta i casi di femminicidio che continuano a verificarsi con un *trend* inarrestabile. Oggi non intervengo per la staffetta ma per esprimere la soddisfazione, mia e delle colleghe del gruppo Articolo 1-Movimento Democratico, per la norma introdotta al codice antimafia che consentirà le misure di prevenzione per gli indiziati di *stalking*. Come è noto, con le modifiche apportate in Aula al Senato è stata ampliata la platea dei reati per i quali sono applicabili le misure di prevenzione. Si è tanto discusso sull'ampliamento ai reati contro la pubblica amministrazione connessi al delitto di associazione a delinquere, che è sicuramente un fatto positivo. Non è però l'unica novità. Nella versione licenziata dal Senato dell'articolo 1 del codice antimafia, che elenca i soggetti destinatari delle misure di prevenzione, sono inclusi anche gli indiziati del delitto di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, cioè il reato di atti persecutori o *stalking*. È una norma molto significativa, che trova fondamento nel dato che si coglie già nella descrizione della fattispecie, che il reato cioè si concretizza quando l'autore compie condotte reiterate. Si tratta, in definitiva di un unico reato che si concretizza in una molteplicità di condotte, ed è perciò un reato abituale. La sua inclusione è perciò perfettamente in linea con la normativa in materia di misure di prevenzione che ne rende possibile l'applicazione in caso di reiterazione di reati o di abitualità. Bene ha fatto, dunque, la Commissione giustizia ad accogliere la proposta del presidente D'Ascola e l'Aula a confermarla. Il punto politicamente più rilevante è che la modifica introdotta nel testo consente di rafforzare sul piano preventivo un argine contro la violenza sulle donne. Questa, considerato il numero di femminicidi che si registrano ogni anno, spesso preceduti da maltrattamenti e violenze di ogni genere, è una necessità perché non può più ignorarsi che i delitti contro le donne hanno bisogno di un serio rafforzamento della sfera. Avremmo voluto anche modificare l'articolo 162-*ter* del codice penale, appena votato in via definitiva alla Camera, per evitare qualsiasi ipotesi di estinzione del reato di *stalking*, ma non è stato possibile. Ho chiesto al presidente D'Ascola di presentare un emendamento in tal senso. Non è però possibile presentare emendamenti che modifichino il codice penale, in quanto materia estranea al codice antimafia. Quindi, l'emendamento sarebbe stato giudicato inammissibile. Comunque sia, la nuova norma introdotta nel codice antimafia, cioè la possibilità di poter sequestrare i beni dello *stalker* in maniera preventiva, segna un serio passo avanti nel contrasto alla violenza sulle donne. Signora Presidente, colleghi, si riporta la notizia, che è di oggi, di un istituto estetico di Asti che cerca una estetista donna che non sia sovrappeso, che possa lavorare undici ore di fila e che non abbia problemi familiari che potrebbero intralciare le prestazioni lavorative. Si cerca, insomma, una donna giovane, magra e sola. Se è pur vero che essere magre e sole talvolta è una scelta fatta in pieno diritto, rispettabile come qualsiasi altra scelta (purché appunto sia legale e civile), è anche vero che risulta amaro che certe caratteristiche finiscano in una offerta di lavoro. lavoro. È comprensibile che un centro estetico e dimagrimento voglia dare la migliore percezione possibile di sé al cliente e che quindi il proprietario o la proprietaria possano privilegiare personale bello, in grado di diventare aspirazionevole per il cliente di rispecchiare quello che in teoria si può fare per lui. Capisco i problemi di comunicazione e *marketing*, la concorrenza e la voglia di fare soldi e successo con la propria impresa. Infatti, io non ce l'ho con questo centro estetico in particolare. Semmai, ritengo che sia proprio il paradigma culturale ad essere finito in una strada oscura, spesso poco dignitosa, soprattutto per la donna. Al di là del fattore estetico che - mi rendo conto - è inevitabilmente qualcosa che cambia la percezione che gli altri hanno di noi (inclusa quella dei datori di lavoro), la parte più difficile da accettare è quella che riguarda la famiglia. Che importanza ha come io riesca ad affrontare in modo efficiente undici ore di lavoro? L'unica cosa che davvero conta è se io ci riesca. Immagino che da parte del datore di lavoro possa esserci la paura che, se uno ha problemi familiari come figli o anziani a carico, una volta firmato il contratto ne possa usare termini e cavilli per essere pagato e strappare qualche ora per l'assistenza o semplicemente quella di ritrovarsi con un dipendente inefficiente. Questo rischio comunque esiste e c'è sempre ovviamente. Le donne hanno grandi capacità di affrontare e gestire più di un problema alla volta, hanno spesso una forza di volontà e una resistenza maggiori di quella maschile e, soprattutto, hanno lo stesso diritto di lavorare e comporre la propria felicità che è riservato agli uomini. Ai maschi però raramente viene chiesto di essere in forma o se hanno bambini o anziani a carico: per lo più si chiede loro competenza e dedizione. Invito tuttavia a riflettere su un punto: se è vero che è una caratteristica specifica della donna quella di restare incinta e partorire, lo è anche la voglia di non annullarsi in quel processo, di dare il meglio di sé e di dimostrare di essere comunque una persona produttiva, competente e presente. Potremmo anche scoprire che, perfino in un centro estetico, anche una donna più grassa e materna può avere un suo valore, magari proprio quel valore che ha raggiunto grazie a dei figli o all'assistenza prestata a degli anziani. Il rischio di smettere di valorizzare la storia delle persone e di concentrarsi su quanto esse efficacemente sanno annullarsi nel lavoro è, sinceramente, un po' pauroso.